Vi era l'accordo tra maggioranza e opposizione di procedere alla votazione, nella seduta che era stata fissata per questa mattina, degli emendamenti al decreto-legge sull'efficienza giudiziaria. Non vi era da parte di nessun componente dell'opposizione alcun atteggiamento ostruzionistico. Tanto per fare un esempio, il Gruppo di Forza Italia non aveva presentato più di 15 o 16 emendamenti.

erano presenti due o tre componenti, mentre si registrava la presenza al completo dei Gruppi di maggioranza. conclusa la fase della illustrazione degli emendamenti, si è disposto di passare alla votazione. Evidentemente una votazione assolutamente inutile, in ragione del fatto che, proprio per l'accordo che vi era stato, vi era l'assenza dei componenti dell'opposizione e la massiccia presenza dei componenti della maggioranza. C'è chi interpreta il proprio ruolo a difesa della maggioranza e dell'opposizione, chi invece interpreta il proprio ruolo appiattendosi sui *desiderata*, anche non accettabili, della maggioranza. Tant'è: non c'è alcun problema. Oggi pomeriggio si passerà ad affrontare questo decreto-legge e quello che si poteva risolvere tranquillamente in Commissione, sarà oggetto di forti discussioni in Aula. Vede, presidente Zanda, quando lei lamenta (come ha fatto una volta), che forse in Commissione si dovrebbe lavorare in maniera diversa per evitare che in Assemblea vi sia un clima di forte tensione, forse dovrebbe fare una riflessione su come vengono condotti i lavori in Commissione.

Orbene, di tutto questo ne parleremo nel pomeriggio, però c'è una cosa che a me preme in maniera particolare. Nel corso della seduta di ieri, avendo il Governo motivato la proroga del pensionamento per sette o otto persone, non di più, sul presupposto che questa proroga era fondamentale per smaltire il rilevante carico di lavoro esistente presso la Cassazione, mi sono permesso di chiedere al rappresentante del Governo di fornirci i dati relativi allo smaltimento delle pendenze a seguito della proroga dell'anno scorso. Infatti se, per ipotesi, nell'anno della precedente proroga non si dovesse registrare un dato apprezzabile in ordine al venir meno delle pendenze, ma le pendenze degli anni precedenti dovessero essere sostanzialmente analoghe all'anno in cui già vi è stata la proroga per un anno di taluni vertici della Cassazione, verrebbe meno il presupposto presupposto esposto dal Governo a fondamento di questo provvedimento. Il Governo si era impegnato a portare questi dati nella seduta, poi sconvocata, di questa mattina della Commissione giustizia. Ho chiamato in Commissione giustizia per sapere se i dati fossero arrivati e ho ricevuto risposta negativa. signor Presidente, ella sa bene come questi dati siano importanti ai fini delle valutazioni che l'Assemblea dovrà assumere con riferimento a questa proroga, perché è evidente che se i dati dovessero dimostrare che la proroga precedente ha avuto esito positivo in ordine all'abbattimento delle pendenze, *nulla quaestio*,

tra l'abbattimento delle pendenze prima della proroga e l'abbattimento delle pendenze nell'anno della proroga, verrebbe meno il presupposto e, venendo meno il presupposto, la norma sostanzialmente si ridurrebbe alla proroga pensionistica di sette Chiedo quindi, signor Presidente, che ella voglia farsi interprete di questa necessità, non solo del Gruppo di Forza Italia ma, immagino, di tutti senatori e chiedere al Governo, per la seduta di oggi pomeriggio, di fornire all'Assemblea i dati che ho richiesto, che sono assolutamente necessari per un corretto convincimento in ordine al voto che dovrà essere espresso sull'articolo 5 del decreto-legge, che oggi esamineremo.*(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la mozione che oggi presentiamo in quest'Aula intendiamo impegnare il Governo a verificare le effettive condizioni di sicurezza nel trasporto dei passeggeri realizzato sull'intera rete in gestione della città di Roma e sulle ferrovie concesse a essa afferenti. Riteniamo infatti che rispetto alle condizioni di una gestione dissennata, aggravata in maniera importante e significativa a partire dagli anni 2010-2011, che avevano portato di fatto l'azienda di trasporto della capitale in una situazione di dissesto economico e finanziario tale da renderne possibile il *default*, le recenti azioni intraprese da parte della nuova Giunta Raggi vedono compromettere anche il faticoso sforzo che era stato precedentemente profuso dalla gestione Rettighieri e Brandolese, insediati con la gestione commissariale del prefetto Tronca. Un breve ma intenso periodo in cui, come abbiamo potuto acclarare anche nel corso di diverse audizioni nella Commissione trasporti di questo Senato, il *management* dell'azienda, a fronte di una situazione ereditata davvero molto grave sotto ogni profilo, aveva intrapreso un difficile e impegnativo percorso di corretta gestione dell'azienda, avviando la ristrutturazione dei servizi di linea che versavano in condizioni disperate, come frequentemente salite agli onori della cronaca anche a livello nazionale. Del resto, Roma non è soltanto una grande e complessa metropoli, difficile da organizzare in termini di mobilità perché anche sede di moltissimi uffici e soggetta ad un pendolarismo di dimensioni e caratteristiche non uguali a nessun'altra realtà italiana. è anche, molto più banalmente, la città più bella al mondo, occasione di visita per decine di milioni di turisti in ogni mese dell'anno e la qualità del trasporto pubblico costituisce, inevitabilmente, il biglietto da visita del nostro Paese. ATAC è da anni un'azienda di trasporto sull'orlo del collasso economico e finanziario grazie ad un debito che si stima si aggiri oggi intorno ad 1,3 miliardi di euro. La situazione in cui versano i mezzi di trasporto nella Capitale, come detto, è il frutto di anni di gestione dissennata, aggravata nel periodo della gestione del sindaco Alemanno da vicende di corruzione e di assunzioni clientelari. Alla complessità ordinaria della gestione si è così aggiunta un'assente o insufficiente manutenzione del parco mezzi, che ha portato a poter disporre di un terzo appena del materiale circolante con conseguenti drastiche soppressioni di corse e disservizi. Ancora oggi l'Azienda ha i più vecchi autobus tra le varie capitali europee con un ciclo di vita ormai superiore agli undici anni, quando sono appena quattro quelli di un autobus a Parigi, cinque quelli a Londra e otto a Madrid. Lo stato di dissesto delle strade ha inciso e incide in maniera non banale sulle condizioni di sollecitazione ai principali organi di funzionamento dei mezzi, con riparazioni più frequenti che nelle altre realtà. Questo comporta la messa fuori servizio di oltre due terzi degli autobus dell'azienda di trasporto pubblico, cui si aggiungono le condizioni inaccettabili di funzionamento del servizio nella tratta ferroviaria Roma-Ostia, per l'utilizzo di treni non adatti a quella tipologia di impiego, ai guasti sull'infrastruttura che, con frequenza crescente dei disservizi, ha visto recentemente e spesso l'utenza abbandonare il mezzo di trasporto e proseguire a piedi in condizioni di assoluta insicurezza. Ed è proprio sul tema sicurezza che la nostra mozione, come ho detto in apertura, vuole soprattutto richiamare l'attenzione del Governo a verificare e vigilare attentamente sulle reali condizioni per la tutela dell'incolumità delle migliaia di persone che ogni giorno prendono i mezzi pubblici di trasporto della città di Roma. Sempre più frequenti sono le notizie di pneumatici deformati o con i battistrada non conformi agli *standard* di circolazione, di ruote e rotaie con difetti di fabbricazione o di mezzi fermi nelle officine di riparazione per l'assenza di pezzi di ricambio, dovuta all'impossibilità di acquisto per la mancanza di fondi, o di mezzi che prendono fuoco per autocombustione. Sappiamo bene che la nuova Giunta si è insediata da pochi mesi e ne ha passati alcuni nel cercare un faticoso assetto che faticherei a definire definitivo, ma è anche vero che i proclami della campagna elettorale facevano attendere risultati ben diversi dal vedere l'attuale assessore vantarsi per l'arrivo di nuovi autobus finanziati ed acquistati, ovviamente, non da questa Giunta. Per questo, signor Presidente, noi chiediamo al Governo di svolgere un'attenta azione di verifica della sicurezza che, ne siamo certi, sarà vista in maniera positiva anche da chi ora è chiamato nei fatti a gestire l'azienda e tutto il complesso sistema del trasporto romano.

sommessamente e modestamente, abbiamo cercato di capire perché da gennaio a oggi vi è circa il 30 per cento di corse in meno,

Il problema dei disservizi del trasporto locale di Roma finisce per travalicare i confini e si pone come un problema di tipo nazionale, data la mole di pendolari, turisti e utenti provenienti da tutta Italia e dal mondo.

giorno dopo giorno si vedono bus fermi, trainati dai carri di soccorso, anche nel centro di Roma, senza parlare delle periferie. Tra un anno, si dice, il 30 per cento dei mezzi sarà da rottamare; non si fa una politica di acquisto di nuovi mezzi e non c'è una politica della mobilità da una decina, quindicina, ventina d'anni a questa parte, responsabili tutte le amministrazioni e i sindaci precedenti e quello attuale che, se il bel tempo si vede dal mattino, sarà una catastrofe per Roma e per i servizi che Roma Capitale dovrebbe fornire. Sommessamente, come Gruppo, chiediamo al Governo di intervenire, affinché il trasporto pubblico della Capitale possa recuperare efficienza e qualità al pari delle altre capitali europee, anche più popolose ed estese (se guardiamo a Parigi e a Londra ci

a stimolare azioni per il potenziamento delle corse e dei mezzi di trasporto di superficie, soprattutto nelle fasce orarie di punta. (**1-00652**) (testo

Mi preme ricordare che, già dal 2014, è stata posta in essere tutta una serie di azioni e di accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi,

del sistema complessivo dell'azienda. Poi ci sono stati la vicenda del commissariamento di Roma e quindi, a cascata, le azioni poste in essere

un altro grave problema, quello della bigliettazione elettronica e dell'elusione. L'amministrazione comunale e l'ATAC incaricarono *pro tempore* il generale della finanza, dottor Rapetto, a svolgere un'analisi puntuale. Ciò è stato fatto e abbiamo chiesto che i risultati venissero resi pubblici, ma l'amministrazione comunale e l'ATAC non li hanno mai tirati fuori.

di presentare un piano nazionale per gli interventi infrastrutturali relativi alla nostra Capitale e di decidere con urgenza

e valuti, anche alla luce delle linee guida in merito alla politica di gestione delle imprese partecipate dalla pubblica amministrazione e degli strumenti di legge attualmente previsti, se sussistano le condizioni per porre in essere una procedura concorsuale, attivando per ATAC un'amministrazione straordinaria speciale. In ultimo, chiediamo al Governo di valutare la possibilità di collocare temporaneamente la partecipazione dell'ATAC all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, affidando contestualmente ad una struttura tecnica scelta *ad hoc* il compito del risanamento industriale e patrimoniale dell'azienda.

al primo posto sta il potenziamento del trasporto pubblico (lo indica 48 per cento degli intervistati). Figuriamoci a Roma, dove la situazione del servizio risulta in costante peggioramento nell'ultimo decennio, con riduzione delle corse e della qualità dell'esercizio, incremento della frequenza di interruzione dei servizi e scadimento costante della manutenzione delle vetture, con i conseguenti rischi in termini di sicurezza per gli utenti, in particolare nelle linee della metropolitana. Alcune tratte, come la Roma-Lido, vincitrice del Premio Caronte, sono diventate il simbolo peggiore del trasporto locale in Italia. Lo scadimento complessivo del servizio marcia di pari passo con la crisi finanziaria e gestionale di ATAC: crescita dell'indebitamento, evasione dagli obblighi tariffari, riduzione del numero di autisti operativi e delle vetture circolanti. Tutto questo nel quadro di una politica di gestione da parte del *management* che ha favorito assunzioni clientelari, irregolarità accertate nella conduzione degli appalti e ritardo nell'operazione di risanamento Secondo le ispezioni condotte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'ANAC la dimensione del danno procurato all'erario e al bilancio di Roma Capitale rileva un debito consolidato che supera gli 1,5 miliardi di euro. Di oltre 1.900 mezzi, 600 sono fermi perché obsoleti. L'esecutivo si è attivato rinviando al 2019 il piano di rientro dell'azienda, ma adesso sono necessarie azioni forti e trasparenti. Il nuovo contratto di servizio 2015-2019 fra Roma Capitale e ATAC sembrerebbe avviarsi sulla china di un procedimento per la riduzione del disavanzo aziendale e l'efficientamento del servizio, la riqualificazione del parco veicoli, l'incremento della produttività e degli investimenti infrastrutturali

ma riteniamo anche che l'Amministrazione capitolina debba fare qualcosa di più delle visite a sorpresa nella sede ATAC, postando foto con l'amministratore unico che afferma «Al lavoro per rilanciare l'azienda». Le operazioni di facciata non bastano, negli anni, anche recenti, ne abbiamo viste continuamente, soprattutto di fronte a scadenze strategiche come quella del 2019, appuntamento con la gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico e dei vincoli per quello su gomma. Per lo sviluppo di una mobilità moderna e sostenibile e il risanamento e la riqualificazione del trasporto pubblico romano servono, oltre alla competenza del *management*, l'impegno sinergico di Roma Capitale, della Regione Lazio, per quanto di competenza anche sul fronte finanziario, e del Governo nazionale che deve manifestare con atti concreti la consapevolezza che si tratta di una sfida decisiva per la Capitale e per la qualità della vita Per questo, nella nostra mozione intendiamo impegnare il Governo a supportare adeguatamente l'azione di risanamento, incrementando la dotazione del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, che vede la Capitale danneggiata nel rapporto *pro capite* risorse-cittadino, a vantaggio di tutte a cominciare dalla stessa Milano. Per necessità di tempo non elencherò gli interventi contenuti nella nostra mozione e in questo mio intervento, che consegnerò agli atti.

il Governo non può parlare di cura del ferro e finanziare costose ed inutili autostrade private come la Tirrenica. La Regione Lazio non può progettare e finanziare l'autostrada Roma-Latina ed abbandonare il ferro esistente ai livelli di degrado attuali e da *record*, come la Roma-Lido e il suo inattaccabile primato, d'Italia. Perché così anche i famosi privati (sempre i soliti noti) che volete coinvolgere scelgono ovviamente le autostrade e su ferro unicamente l'Alta Velocità (la polpa). Ogni giorno centinaia di migliaia di automobili convergono su Roma: è assurdo, è sbagliato, è costoso, è, dal punto di vista ambientale, catastrofico. Linee Roma-Viterbo, Roma-Lido, Roma-Latina; e chiusura dell'anello ferroviario; ferro di superficie e/o e/o sopraelevato, soprattutto nelle medie ed estreme periferie, molto meno costoso e con gli stessi *standard* di velocità; su gomma, mezzi elettrici o ibridi: queste sono le scelte di campo, il patto che gli attori della politica devono stipulare. Sarebbe per Roma un'assoluta rivoluzione. Credo che su questo ci dobbiamo sfidare e su questo, non sulla pratica delle assunzioni clientelari

Signor Presidente, parlare di trasporto pubblico locale nel nostro Paese non è facile, perché partiamo dal dato oggettivo per cui siamo il fanalino di coda in Europa. Se poi dobbiamo parlare del trasporto

degli ultimi quindici anni, la maggior parte dei finanziamenti da parte dei Governi che si sono succeduti è stata erogata quasi esclusivamente per l'alta velocità. Di fatto,

tali contesti abbiamo comunque delle situazioni se non di eccellenza, comunque potabilissime: questi sono dati scientifici, che tutti possono consultare. È chiaro che risulta difficile parlare di TPL quando da un Governo come quello attuale viene la proposta di una possibile fusione tra ANAS e

sarà abbastanza difficile capirlo. Ci sono dei dati incontrovertibili dal punto di vista delle analisi che bisogna fare, per capire il trasporto pubblico nel nostro Paese è bene citarli. Per quanto riguarda i chilometri effettivi di metropolitane e ferrovie suburbane, Milano è la città

Roma all'ultimo posto per quanto riguarda il trasporto pubblico locale in ambito europeo. Chiediamo dunque al Governo non di cambiare dalla sera alla mattina lo stato delle cose, ma di cominciare a piccoli passi.

disponendo che l'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico andasse determinato tenendo conto, oltre che dei costi *standard*, anche della fornitura di un livello adeguato del servizio. Pertanto, chiediamo al Governo di mettere in atto dei provvedimenti normativi affinché si proceda a una ripartizione dei finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale sulla base dei fabbisogni e dei costi *standard*, al fine di premiare gli enti che riescono a erogare il servizio a costi minori,

Signor Presidente, parlare della mobilità di Roma è sempre particolarmente interessante, perché va ricordato che questa città ha la più alta percentuale di automobili per numero di abitanti in Europa, esistendo 710 automobili per ogni 1.000 abitanti. Il numero dei veicoli circolanti a Roma è di circa 930

L'approccio che la Giunta sta provando ad attuare è immaginare un percorso diverso, in cui i mezzi siano effettivamente

perché trasferisce al servizio pubblico locale romano una quota inferiore a quella che gli dovrebbe

si è evoluta nel corso degli anni fino ad arrivare a quella attuale, che vede l'ATAC con un debito pregresso di 1.400 milioni di euro.

che sono stati stranamente spostati dal commissario Tronca; c'erano 58 milioni a disposizione dell'ATAC per interventi che sembravano utili e stranamente il commissario Tronca li ha fatti sparire. Si

bisogna revisionare le testate, bisogna farli andare. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Per non parlare della Roma-Ostia,

il Governo deve aiutare la Giunta a far sì che i cittadini romani, che rappresentano i cittadini della Capitale d'Italia, abbiano un servizio adeguato a quello che dev'essere loro offerto. offerto. Lo scopo che dobbiamo raggiungere è dare il servizio ai cittadini. Non pensate che aver lasciato ATAC in questo modo ci scoraggi. Noi non ci scoraggiamo, e daremo ai cittadini quel servizio di cui hanno bisogno. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, dai senatori Filippi, Aracri ed altri. Conseguentemente sono state ritirate le mozioni nn. 619 e 653.

sono ormai venti-trent'anni che il trasporto pubblico a Roma non funziona. Per questo voglio esporre e depositare i dati di Trambus fino al 2008. Trambus è la società che gestiva il servizio pubblico romano. Dal 2000 al 2008 ha avuto un risparmio di circa 1.000 persone. Nel 2008 i chilometri erogati da Trambus erano 116 milioni, contro i 90 milioni di oggi. Il risparmio è stato, dal 2000 al 2008, di 478 milioni per il costo del personale. I non idonei, cioè coloro che non volevano più guidare ma andare negli uffici, sono il personale non alla guida nel 2008 si riduce al 25 per cento contro il 32 per cento del 2000 (il che vuol dire più autisti). La verità nel nostro Paese va ristabilita, Presidente, altrimenti anche le buone esperienze vengono travolte dal più bieco populismo, e questo non è più accettabile. Le chiedo il testo integrale del mio intervento, che è molto più ampio, affinché questa verità venga ristabilita e affinché tutte quelle che sono state le buone pratiche che si sono svolte in questa città abbiano finalmente la possibilità di essere riconosciute per quelle che sono state.

che le competenze in materia di amministrazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono poste in capo alla Regione competente per territorio, ovvero per delega all'ente locale competente, e che le competenze gestionali di ATAC sono in capo all'organo di amministrazione della medesima società e, indirettamente, possono riferirsi al socio Roma Capitale. Certamente il miglioramento della mobilità dei cittadini dentro le aree urbane rappresenta l'obiettivo di chi governa le istituzioni. Infatti, il trasporto pubblico locale, anche nella sinergia che definiamo che definiamo per semplicità ferro-gomma, è l'unica vera soluzione strutturale per risolvere il problema di inquinamento e congestione delle città. A questo fine il Governo ha da tempo messo in campo alcune azioni. Mi riferisco innanzitutto al decreto legislativo sui servizi pubblici locali, sul quale in questi giorni le competenti Commissioni di Camera e Senato stanno per esprimere il loro parere. Il Governo, inoltre, in attuazione della normativa vigente sta già operando verso un sistema che preveda l'adozione dei costi *standard*; infatti, un decreto ministeriale ha già ottenuto il parere favorevole in sede tecnica da parte della Conferenza unificata e si è in attesa del parere politico. Segnalo, poi, il rinnovo del parco rotabile: infatti, il parco autobus italiano viaggia con una vita media di circa dodici anni rispetto ai circa otto anni di vita media in Europa; da qui un investimento massiccio di risorse per rinnovare il parco bus, soprattutto nelle città. Ricordo che sono stati già trasferiti 350 milioni di euro alle regioni per l'acquisto di nuovi autobus, mentre altri 150 milioni sono pronti per essere trasferiti nel corso del prossimo anno. ciò, abbiamo stanziato circa 640 milioni per il rinnovo del parco rotabile in campo ferroviario. Per quanto attiene, invece, alla materia della sicurezza dei servizi di trasporto ad impianti fissi, essa residua in capo all'amministrazione centrale ovvero, per i servizi eserciti sulle ferrovie interconnesse, in capo all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle In particolare, la vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, per i servizi di trasporto pubblico sull'intera rete ad impianti fissi delle ferrovie concesse,

Proprio in tale ambito, a seguito di una serie di reiterati malfunzionamenti sulle linee ferroviarie e metropolitane, la citata direzione generale ha istituito una commissione interministeriale appositamente dedicata ad implementare il monitoraggio sul processo di gestione della sicurezza delle linee medesime messo a punto dalla società ATAC. La commissione ha in corso una complessa attività istruttoria che comprende sia l'esame di materiale documentale che l'espletamento di specifiche ispezioni *in loco*. Inoltre, nell'ambito del più ampio processo nazionale di implementazione della sicurezza dei servizi ferroviari, sono state destinate ad interventi in materia di sicurezza presso le ferrovie in concessione o rientranti nella ex gestione commissariale governativa,

soltanto delle parti dispositive modificate, evitando di leggere i cinque capoversi che sono rimasti immutati. Le parti dispositive modificate sono gli ultimi due periodi. come segue: «a valutare, anche alla luce delle linee guida governative in merito alla politica di gestione delle imprese partecipate dalla pubblica amministrazione ed agli strumenti di legge previsti, se sussistano le condizioni per porre in essere procedure idonee a sostenere il rilancio dell'azienda anche attraverso procedure

di un organismo statale dotato delle necessarie competenze, affidando contestualmente ad una struttura tecnica scelta *ad hoc* il compito del risanamento industriale e patrimoniale dell'azienda». Queste sono le due parti dispositive riformulate.

mi permetto di suggerire la seguente riformulazione: «impegna il Governo a favorire il miglioramento del trasporto pubblico locale, dando attuazione al decreto legislativo sui servizi pubblici locali in corso di emanazione». «per quanto di competenza, a intervenire affinché sia garantita la sicurezza di passeggeri e personale in tutti i mezzi di trasporto pubblico circolanti a Roma». Il terzo punto del dispositivo non è di nostra competenza e, quindi, si chiede di cassarlo.

il triennio 2017-2019, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, «a prevedere adeguata dotazione finanziaria, nei limiti delle disponibilità di settore, per gli investimenti contenuti nel programma delle infrastrutture strategiche si impegna il Governo «nell'ambito delle proprie competenze, a monitorare, per il tramite degli organi di controllo, le condizioni di esercizio e sicurezza della rete del trasporto pubblico di Roma, con riferimento particolare allo stato delle linee della metropolitana, a tutela della sicurezza degli utenti e del personale addetto».

punto del dispositivo si impegna il Governo «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di incrementare nel triennio 2017-2019 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico

che assegnerà al vincitore - a chi sarà in grado di vincere la gara - la gestione del trasporto pubblico romano. Una gara di queste dimensioni, colleghi senatori - e mi rivolgo anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che oggi si trovano ad amministrare la città di fatto vedrà l'amministrazione tra pochissimo già impegnata perché, per averla già aggiudicata entro il 31 dicembre 2018, è ovvio che le procedure dovranno partire addirittura dalla seconda metà del 2017.

Ancora non è chiaro se il debito precedente verrà o no garantito - è stato fatto prima - con l'appostamento di una serie di operazioni che riguardano il patrimonio dell'ATAC a garanzia di quel debito. Qualora venisse meno questa condizione, probabilmente l'ATAC andrebbe direttamente con i libri in tribunale. Ci è quindi sembrato - è sembrato a me, al collega Aracri e a molti altri che hanno lavorato in questa giornata - che l'occasione fosse utile per evitare di fare polemiche e cronistorie varie sulla storia dell'ATAC,

come mettere sul tappeto delle procedure che consentano al Governo, da un lato, e all'amministrazione comunale, dall'altro, di trovare se non un punto di incontro, per lo meno una via di uscita a questa situazione che a me pare molto, ma molto trascinata in avanti e molto prossima ad arrivare al punto di non ritorno. Da questo punto di vista, il prodotto finale è stato l'ordine del giorno in esame, su cui ci siamo incontrati con i colleghi del Partito Democratico, che rimette la palla anche nel campo del Governo

che sia sufficiente strangolare definitivamente l'ATAC nei prossimi diciotto mesi giocando a un rimpallo di responsabilità per aprire la strada a qualcuno che poi parte già avvantaggiato nella gara, deve sapere che anche fuori da quest'Aula si vigilerà perché ciò non accada.

ci si dovrebbe solo vergognare per quello a cui abbiamo assistito nel corso degli anni nella gestione del trasporto pubblico romano.

tentando di creare all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze una *bad company* dove catapultare ATAC e tutte le sue porcate, cercando di ripulirla e ripianarla. Ci aspettavamo che una mozione presentata in Senato potesse avere il valore di indicare indicare alla politica nazionale il principio che deve ispirare la programmazione e la realizzazione del sistema trasportistico di una metropoli moderna. moderna. Signor Vice Ministro, ci sono tutti gli ingredienti: basta saperli usare e cucinare, all'interno delle direttive - e non solo - che ci dà la Commissione europea.

Noi alziamo le mani perché non abbiamo responsabilità dirette. A mio avviso, però, qualcuno dovrebbe vergognarsi questa mattina. Nel mio intervento precedente ho ricordato che il trasporto pubblico locale viene realizzato con grandi sacrifici anche al di fuori delle metropoli,

In una metropoli è solo una questione di organizzazione, e non lo dico io ma chi ne sa più di me: lo dice la Commissione europea. Il tentativo di stamattina mi lascia un po' l'amaro in bocca, e lo dico sinceramente. Noi ci asterremo perché sicuramente è una questione all'interno della quale non vogliamo entrare, essendo molto articolata, e non perché non vogliamo assumerci le nostre responsabilità. Ma la questione non si risolve sicuramente con questo tentativo. sicuramente con questo tentativo. Mi dispiace, cari colleghi, e lo dico anche a chi è stato solido amministratore. Vedo il collega Albertini, che è stato sindaco di Milano: non avrebbe mai fatto una cosa del genere! Oggi anche lui, come me, arrossirebbe e probabilmente si vergognerebbe a dovere sottostare a determinate questioni e regole politiche. Purtroppo, questo questo è il trasporto pubblico romano e ne siamo tutti consapevoli. Noi ci asterremo, arrangiatevi, affari vostri! Non c'entriamo nulla.

su come articolare l'azione di risanamento, impegnando il Governo a fare quello che sarebbe doveroso fare per la propria Capitale, e cioè supportare

assolutamente oscuro - forse bisognerebbe dire le cose come sono - che va nel tentativo di avocare centralmente la gestione dell'ATAC. Chi presenta questo ordine del giorno? Lo presenta il senatore Stefano

già il fatto che oggi discutiamo di una mozione sull'ATAC mi sembra alquanto singolare. Ma ci sta. Da tre mesi

Ricordiamo che avete governato diciassette anni. E il diciassette dalle mie parti porta sfortuna. Ma non ha portato sfortuna a voi. Ha portato sfortuna ai cittadini romani, che sono quelli che pagano il fio delle vostre malefatte. Voi siete quelli di Mafia Capitale. Non dimentichiamolo mai!

Voi siete quelli che avevano tra le loro fila il marito della signora di cui abbiamo parlato prima, che è l'assessore con la casa in Campidoglio, condannato a due anni e due mesi per corruzione. Potremmo parlare anche di Luca Odevaine, il facilitatore di Buzzi, che era il vice capo di gabinetto di Veltroni: due anni e due mesi, 250.000 euro di mazzette da restituire. Potemmo fare una lunga lista, ma consolatevi, amici del PD,

per questo - senza che ci sia una valutazione che naturalmente riguarderà la storia e, quindi, anche le amministrazioni che hanno governato questa Città, anche se noi siamo certi che la tradizione di

qualcuno che non sia diverso dal Partito Democratico. Se Cantone ha potuto certificare che gli appalti in quella azienda negli ultimi cinque anni sono stati fuori regola, lo si deve al fatto che qualcuno ha aperto dei cassetti. senatore Cioffi, le consiglieri di suggerire all'amministrazione che lei sostiene di non tornare indietro su questo, perché gli atti di questi tre mesi certificano esattamente il contrario, cioè che tutti quelli che in quell'azienda hanno aperto i cassetti li avete presi e li avete mandati a casa. Voi li avete mandati a casa, caro senatore Cioffi, e li avete sostituiti con parenti

Quindi, caro senatore Cioffi, tutte le strade per evitare che quell'azienda, vista la strategia che avete messo in campo, compresa quella di non valorizzare il patrimonio che ha quell'azienda...*(Proteste

Senatore Aracri, lei non ha fatto una dichiarazione di voto, dunque si intende che, dopo il ritiro della sua mozione, condivida la stesura dell'ordine del giorno G1, così come riformulato. Colleghi, prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.